sono qui a riferire sugli eventi che hanno causato la tragica morte di quattro militari ed il ferimento di un altro soldato del nostro contingente in Afghanistan. La ringrazio, Presidente, per avermi dato la parola e ringrazio altresì i colleghi presenti. Sento il dovere, innanzitutto, di esprimere il più sincero e profondo cordoglio alle famiglie dei giovani militari deceduti e la vicinanza al militare ferito, cui va l'augurio di un pronto ristabilimento. Abbiamo, ancora una volta, purtroppo, in un'occasione drammatica, la tragica prova dello spessore del coraggio che spinge tanti ragazzi ad arruolarsi nelle Forze armate. Quel coraggio che rende possibile l'affermazione della pace, della libertà, nella democrazia, in territori geograficamente remoti, ma determinanti per le sorti della nostra civiltà. Oggi rendiamo loro un omaggio sincero e profondo, con il dolore nel cuore e con il senso pieno di una responsabilità che rendono questo passaggio parlamentare tutt'altro che rituale. Sono certo che questa Aula è unita nell'espressione di questi sentimenti. Signor Presidente, onorevoli senatori, fatta questa doverosa e sentita premessa, passo a descrivere i fatti secondo la ricostruzione effettuata sulla base delle notizie finora pervenute, ricordando che, come sempre in queste occasioni, una squadra di Carabinieri è sul posto, ancora ora, per tutti gli accertamenti tecnici e scientifici che possono meglio determinare le circostanze in cui l'evento si è determinato. Il quadro in cui si inserisce tale evento è caratterizzato da una continua evoluzione operativa. Nell'ambito dei compiti assegnati al nostro contingente, a partire dal 1° settembre di quest'anno, la *Task Force South East*, che fa parte del *Regional Command* *West* a guida italiana, ha assunto la responsabilità dei distretti di Bakwa, Golestan e Por Chaman della provincia di Farah, operando dalle basi di Bakwa, Buji e Golestan.

zona Ovest era stata temporaneamente assegnata al controllo degli Stati Uniti ed è tornata da poco sotto il controllo italiano. Tale controllo è stato assegnato al 7° Reggimento Alpini, il cui personale ha iniziato ad affluire in teatro nella seconda metà del mese di luglio per familiarizzare con le procedure operative e con il territorio. La principale attività è rivolta al controllo del territorio lungo gli itinerari più importanti, al fine di garantire la libertà di movimento alle forze amiche e alla popolazione. Il 9 ottobre 2010, alle ore 9,35 locali (7,05 ora italiana), un reparto nazionale è stato ingaggiato da forze ostili con fuoco di armi leggere e lanciarazzi controcarro a 1,5 km a Nord Est dalla base di Buji. L'unità, del livello di compagnia, era costituita da circa 120 uomini su 38 mezzi (34 VTLM Lince e 4 mezzi speciali del genio), per la gran parte dotati di dispositivi di disturbo elettronico (i cosiddetti *jammers*), detto - alla *Task Force* *South East* su base 7° Reggimento Alpini di Belluno, che scortavano un convoglio di rifornimenti logistici di 74 mezzi civili guidati da autisti locali, che precedentemente avevano rifornito le nostre basi nell'area. Al momento dell'attacco, condotto da un nucleo presumibilmente di una trentina di *insurgents,* il convoglio stava muovendo lungo una pista ricavata nell'alveo di un torrente asciutto, parallelo alla strada, per diversificare l'itinerario di spostamento.

dall'esplosione che ha causato il decesso di quattro occupanti e il ferimento di un quinto. Le nostre unità hanno immediatamente risposto al fuoco con un'intensa reazione, durata 30-40 minuti, che ha disperso gli *insurgents*. Per meglio precisare, l'esplosione è intervenuta durante il conflitto, tanto che il nostro mezzo aveva dovuto fare retromarcia perché sottoposto al fuoco degli *insurgents*. Nell'azione sono intervenuti due aerei F16 americani, che hanno effettuato azione di fuoco contro gli *insurgents* impiegando la mitragliera di bordo. Durante lo scontro alcuni mezzi civili del convoglio sono stati abbandonati

per assicurare assistenza sanitaria e per effettuare i rilievi del caso. Sullo stesso itinerario, ma sulla strada e non sulla pista del torrente, nelle giornate precedenti due mezzi del genio, uno statunitense e uno italiano, erano rimasti coinvolti nell'esplosione di due ordigni esplosivi improvvisati, che avevano però fortunatamente provocato danni soltanto ai mezzi e non alle persone.

il caporal maggiore Marco Pedone: tutti celibi ed effettivi al 7° Reggimento Alpini di Belluno. I primi tre avevano già svolto missioni in teatri operativi e avevano una lunga esperienza professionale. Per il caporal maggiore Pedone si trattava invece della prima missione. Nell'azione è rimasto ferito anche il caporal maggiore scelto Luca Cornacchia, dell'Aquila, anch'egli effettivo al 7° Reggimento Alpini di Belluno, coniugato e residente a Lecce Inizialmente trasportato all'ospedale da campo di Delaram e successivamente trasferito a quello di Camp Dwyer, entrambi statunitensi, è stato sottoposto a TAC, che ha evidenziato una frattura di due vertebre lombari, una sospetta contusione polmonare, una frattura al piede destro e lesioni multifocali alla milza. Al momento, le sue condizioni risultano stabili, non gravi, e viene tenuto ovviamente sotto osservazione. Questa mattina è stato trasferito all'ospedale da campo della nostra base di Herat e sarà trasportato in Patria appena possibile. Durante la notte tra il 9 e il 10 ottobre, successivamente allo scontro, il convoglio ha sostato nella base di Buji per riorganizzare il dispositivo e ripianare le scorte. alle ore 8 locali (5,30 ora italiana), durante la prosecuzione del movimento verso Delaram, il convoglio ha subito un ulteriore attacco da parte di un gruppo di *insurgents* con fuoco di armi leggere e lanciarazzi controcarri. Le nostre unità, supportate da due aerei Mirage 2000 francesi e due elicotteri italiani, hanno prontamente risposto al fuoco e si sono sganciati senza danni a mezzi o personale italiano, proseguendo il movimento e completando la missione di scorta. Ricordo che nell'episodio luttuoso è rimasto ferito anche un civile afgano, che era alla guida di uno dei mezzi. Signor Presidente, onorevoli senatori, questa è la ricostruzione dell'evento che ha visto ancora una volta coinvolto un veicolo Lince. Come ho più volte ripetuto, si tratta di un blindato concepito allo stato dell'arte tecnologico e progettuale nel settore della protezione balistica ed antimina. In campo mondiale, al momento, tra i veicoli della stessa categoria è il migliore: non risulta disponibile un'alternativa che possa garantire livelli di protezione del personale superiori. nell'ambito delle misure tese al miglioramento della sicurezza del personale, sono stati già immessi nel teatro afgano 17 esemplari di veicolo blindato medio Freccia, che sono operativi già dal mese di agosto. È bene ricordare che il Freccia è destinato non a sostituire, ma ad integrare gli attuali assetti operativi basati sul Lince, trattandosi di due tipi di veicoli in grado di operare in modo complementare. Vorrei precisare che ciascun elemento protettivo e difensivo ha sempre un limite in risposta alla minaccia: se cresce la minaccia, si provvede con nuovi sistemi di difesa, in una sorta di *loop* *in* *escalation* che ricalca lo schema storicamente provato della cosiddetta contrapposizione lancia-scudo o proiettile-corazza. Per tale ragione non si possono considerare risolutive le soluzioni tecnico-costruttive rispetto alle minacce del tipo in questione. Quello che risulta fondamentale è, invece, il sistema complessivo posto in atto per fronteggiare la minaccia, nel cui ambito, oltre alla protezione dei mezzi, rientrano l*'intelligence*, la ricognizione aerea delle rotte terrestri mediante velivoli senza pilota (i cosiddetti Predator), il supporto aereo, le tattiche di movimento, le tecniche di osservazione del terreno, l'addestramento del personale e anche le interrelazioni con la popolazione locale. Tutti questi elementi costituiscono il sistema complessivo che consente di fronteggiare una minaccia; ma è evidente che non esiste nessun sistema per eliminare il pericolo in condizioni quelle che sono presenti in qualunque missione, anche di pace, il cui presupposto è comunque la possibilità di uso legittimo della forza giusta. Signor Presidente, onorevoli senatori, due sono le questioni

in uso e nella disponibilità del nostro contingente, o comunque del contingente internazionale, e quella inerente la durata della missione in Afghanistan. Pur in un'occasione in cui è prevalente il compito di riferire

della nostra missione in Afghanistan sono e rimangono quelli definiti e condivisi in ambito Alleanza Atlantica e sottoposti all'avallo del Parlamento: circa la natura della missione,

dal desiderio di affermare la realtà, qualche altra volta un po' strumentale, sulla natura costituzionale della nostra missione in Afghanistan, detto e ribadito che essa si pone

Ricordo che questo termine viene usato, in fase di comunicazione, in mille le occasioni: la guerra alla mafia, la guerra alla camorra, la guerra alla droga, la guerra di vista terminologico, la nostra missione di pace comporta atti che, in termini di comunicazione, possono essere definiti di di guerra, così come voi stessi avete definito l'azione di contrapposizione alla criminalità organizzata in varie parti del nostro stesso Paese; figurarsi dunque se non possono essere definiti come di guerra atti di uso della forza giusta e legittima in un territorio in cui le minacce al nostro contingente sono decisive. La questione tuttavia non è terminologica, ma è se la missione risponde o contravviene al nostro dettato costituzionale. Non ci sarebbe bisogno che mi soffermassi più di un secondo su questo problema, avendolo risolto - e mi inchino alle sue parole - in maniera lapidaria, vorrei dire, e, comunque, serena e definitiva ieri (non un anno fa) il Presidente della Repubblica, citando in un suo comunicato ufficiale la rispondenza al dettato dell'articolo 11 della nostra Costituzione della missione internazionale. Io posso solo dire cosa non è

non rientra in alcuna di queste ipotesi: non siamo andati in Afghanistan per conculcare la libertà dell'Afghanistan;

chiarisce in maniera cristallina che vi può essere una limitazione alla sovranità per «un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» e che addirittura l'Italia «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Vi ho detto che cosa non è la nostra missione; vi dico che cosa è: è un'azione per promuovere la pace e la giustizia sotto l'egida di un'organizzazione internazionale. Continuare ad insistere su questo tema, specie dopo le parole del Presidente della Repubblica, mi sembra un esercizio teso a confondere, e che non appartiene alla comune volontà, che riconosco all'intero Parlamento, di affrontare la questione in maniera seria, in maniera seria, determinata e leale, avendo sempre di mira gli interessi nazionali, gli interessi della comunità internazionale ed anche la sicurezza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze in divisa. divisa. I due problemi quindi sono la dotazione dei mezzi e delle armi e la durata della missione. le armi ed i mezzi che possono assicurare un *plus* di sicurezza ai nostri militari. Ho citato i Freccia: potrei ricordare le ralle, cioè le torrette che abbiamo voluto fossero prontamente installate, ed i *jammers*, cioè i dissuasori elettronici di cui abbiamo voluto cui abbiamo voluto fossero dotati tutti i mezzi. Potrei parlare del raddoppio del numero degli elicotteri da combattimento e dell'aumento considerevole degli elicotteri da trasporto: il numero degli elicotteri non basta mai, e mi auguro di poterlo ancora aumentare, e difatti altri tre elicotteri sono pronti a partire. Potrei andare avanti con la qualità dell'addestramento. Abbiamo inviato in teatro prima i Tornado e poi gli AMX, cioè degli aerei. Per che cosa? Per offrire ai nostri soldati, ove fosse necessario, un *plus* di sicurezza quando fossero attaccati. Con orgoglio credo che il mio orgoglio sia il vostro orgoglio - posso affermare che in alcun caso, nei nove anni in cui siamo stati in Afghanistan ed anche nelle altre missioni internazionali, mai un soldato italiano ha dato adito ad alcun tipo di osservazione circa l'impiego delle armi; intendo dire che mai un soldato italiano è andato oltre il legittimo e necessario uso delle armi e mai ha provocato danni ai civili. danni ai civili. È un orgoglio che appartiene al nostro modo di intendere la nostra presenza nelle missioni internazionali, senza per questo volerlo confrontare o paragonare con quello di altri Stati, anch'essi, immagino, spinti dallo stesso desiderio, ma forse a volte con diverse sensibilità. È chiaro, l'ho detto poc'anzi, che all'innalzarsi delle minacce corrisponde un aumento dei mezzi di sicurezza, ma anche che, viceversa, più aumentiamo i mezzi di sicurezza più le minacce sono alte. Ne è la riprova l'entità dell'esplosivo messo in campo in quest'ultima occasione, esplosivo che doveva essere potentissimo se è vero che, in tante altre occasioni, i Lince hanno salvato vite umane rendendo inutili le esplosioni, tanto da essere definiti dai nostri soldati «San Lince» e tanto da essere stati acquistati da contingenti stranieri, quali quello inglese. Si è aperto il dibattito sull'opportunità o meno di dotare del completo armamento gli AMX, cioè gli aerei che abbiamo schierato in teatro. Voglio premettere che non si tratterebbe di una modifica

con le modalità che hanno ritenuto necessarie. Non si tratta, quindi, di assicurare una sicurezza che altrimenti non c'è, né di modificare il comportamento dei nostri militari, che cambia poco, anche in diritto. Se agiscono direttamente con nostri aerei o se li richiamano perché questi operino, non cambia assolutamente nulla. Abbiamo sottoposto a voi, in termini di dibattito e non di decisione, l'opportunità di inviare l'armamento ai nostri aerei, perché i nostri militari,

decisione, che in quel contesto tattico, che i militari mi avevano lealmente e correttamente illustrato, in cui si operava soprattutto in aree a forte densità abitativa,

fase - i comandi NATO avevano dato direttive, come noi desideravamo, assai stringenti e assai limitative sul loro uso, proprio per evitare il rischio di colpire obiettivi non voluti - fosse più

i militari quella opportunità in una mutata condizione tattica, in cui si opera prevalentemente in zone desertiche e con mutate regole di impiego degli armamenti disposte dal comando, non me la sono sentita di dire subito sì alla loro richiesta senza aver prima ottenuto, non un voto, non una decisione, ma un'opinione, per me importante non ho detto del Parlamento - delle Commissioni parlamentari. Ribadisco questa opportunità: potrà avvenire nelle Commissioni; può avvenire anche fuori da esse qualora mi rendessi conto che l'occasione di un dibattito al loro interno servirebbe

un grande vantaggio che abbiamo: quello della condivisione molto larga delle ragioni che ci inducono a perseverare nella nostra presenza in Afghanistan. Io considero uno dei grandi risultati del Parlamento essere riusciti, addirittura una volta senza neanche un voto contrario alla Camera, a votare in maniera comune e positiva i rifinanziamenti delle missioni internazionali. Non sono disposto a mettere a rischio questo spirito comune di sostegno ai nostri militari, che so che vale per loro più di dieci bombe, più di dieci Lince, più di tante altre cose. Mi riferisco al sostegno della Patria, della Nazione, degli italiani, del Parlamento

la decisione che prenderò sarà però non soltanto in funzione tecnica, ma anche con lo sguardo a quest'altro elemento che vi ho appena illustrato, ritenendo così non di fare un piacere ad una parte politica o alla serenità del Parlamento, Parlamento, ma di fare il bene dei nostri militari, che chiedono e sentono come necessario l'appoggio di tutta la comunità nazionale. Lo verificheremo anche dai vostri interventi oggi o dal dibattito che proseguirà. L'altro tema è quello della durata della missione. La missione fino a due anni fa è stata caratterizzata da modalità assai diverse da quelle attuali. Non ho timore di affermare, magari esagerando che, se le modalità fossero rimaste quelle, il tempo di permanenza in Afghanistan della missione internazionale avrebbe potuto essere considerato infinito o indeterminato, salvo un rientro che avrebbe reso inutile il tempo di permanenza passato in quel posto. Non che fosse inutile la presenza, ma non era una strategia che potesse portare ad una risoluzione della questione.

dei nemici della democrazia e della libertà. Questo ha consentito, però, che nel frattempo crescesse in Afghanistan la possibilità di dar vita ad un Governo democratico. Nel frattempo, nelle zone dove comunque questa prima parte dell'operazione si è compiuta, oltre alla presenza militare, abbiamo realizzato 90 progetti riferiti all'educazione, tra cui la costruzione di 50 scuole; 63 progetti relativi alla salute, fra cui la costruzione di ambulatori sanitari, forniture di attrezzatura e farmaci (mi riferisco ad operazioni fatte solo dal contingente italiano), operazioni nel sociale, con 130 progetti relativi alle reti idriche, alla realizzazione di centri per mutilati e disabili, al sostegno della condizione femminile; 90 progetti relativi alla fornitura di materiale per il funzionamento degli uffici governativi e della forza di polizia; 89 progetti riferiti all'agricoltura, relativi alla realizzazione di pozzi per l'irrigazione e di strade rurali e alla fornitura di oltre 50 tonnellate di bulbi di zafferano per la riconversione, in alcune zone nostre già realizzata, dalla coltura del papavero a quella appunto dello zafferano. Tutto questo rappresenta uno dei veri oggetti della presenza, forse per gli afgani sicuramente più importante, ed ancora più lo rappresenta la crescita della democrazia in quel Paese, con tutto ciò che avete già sentito rispetto alla condizione femminile alla possibilità di crescita. L'altro elemento determinante, anche nei primi anni, è stato quello di tenere il più lontano possibile dalle nostre città, dalle nostre famiglie, dalle nostre case, il pericolo del terrorismo: che è la ragione prima per cui siamo andati e restiamo in Afghanistan, la ragione che ci ha indotto a scendere in campo insieme alle altre Nazioni. Quanto essa è connessa alla strategia di questi due ultimi anni. In questi due ultimi anni la strategia è mutata: si è passati da una fase di presidio, per consentire la crescita che ho appena descritto, ad una volontà di controllare effettivamente il territorio per poter fissare un orizzonte temporale entro il quale consegnare al legittimo Governo afgano il compito di governare realmente, con le proprie Forze armate, con le proprie forze di polizia. Non abbiamo alcuna speranza, intenzione o volontà di trasformare l'Afghanistan nella Svizzera. A volte vedo l'elenco delle cose che non funzionano in Afghanistan. Non vorrei che qualcuno prima o poi facesse l'elenco delle cose che non funzionano in Italia, in Francia, in Germania; molto minori, naturalmente, ma che ci sono e ci saranno. Figurarsi in Afghanistan: ce ne saranno sempre. Il nostro obiettivo è quello di consegnare al legittimo Governo afgano un territorio sufficientemente controllato, di modo che tocchi a loro contrapporsi al terrorismo, ai signori della guerra, ai signori della droga. Questo comporta un accrescimento notevole della nostra presenza e dell'azione del contingente internazionale, in particolare anche del nostro contingente. Questa azione - vi prego di attenzionare questo elemento - non è ipotetica; ha già prodotto frutti concreti. Abbiamo già riconsegnato al Governo regionale afgano di Herat il territorio di quella città e della zona circonvicina: lì abbiamo in sostanza già terminato il nostro compito operativo. Io ho la speranza (sempre in accordo con gli organismi internazionali, sempre in accordo con il comando ISAF, sempre in accordo con la NATO) di poter far sì che l'Italia nella zona di sua competenza - la zona Ovest, larga come il Settentrione d'Italia - possa prima che in altre zone completare quest'opera, consegnare ai Governi regionali e al Governo legittimo nazionale un territorio sufficientemente controllato, di modo che tocchi a loro, e solo a loro, il compito operativo. Quando avverrà questo? Vi sono concrete possibilità - se opereremo in concordia,

possa essere consegnata all'Afghanistan legittimo entro la fine del 2011. Significa che a quel punto la nostra missione sarà finita? No: l'arco temporale di cui ha parlato Obama è il 2013, qualcuno è andato addirittura di qualche mese oltre, ma io penso che l'Italia possa ragionevolmente sperare che in larghissima parte del territorio dell'Ovest entro il 2011 le nostre funzioni possano diventare solo quelle di addestramento delle Forze armate e della Polizia. Certo, bisognerà discutere (e lo faremo con Petraeus che verrà qui la settimana prossima; lo faremo a Bruxelles, dove andremo domani; lo faremo a Lisbona nel mese prossimo) sugli assetti successivi al graduale ritengo che noi si debba comunque restare come *combat* nella nostra zona, e sarà la tesi che il Governo italiano dovrà cercare, in amicizia ma nel confronto, di affermare nelle sedi internazionali, di modo che a maggiori risultati corrisponda non una diminuzione

una eccellenza assoluta, sicuramente per quanto riguarda le forze di polizia, per la specificità dei nostri Carabinieri, ma anche dei nostri ufficiali delle Forze armate, in grado di addestrare come pochi come pochi - i militari afgani, perché a loro insegnano non soltanto a combattere, ma insegnano quel modo tutto italiano di rapportarsi con le popolazioni civili che ha contraddistinto da sempre la nostra presenza nelle missioni internazionali. Ho cercato di darvi degli elementi, e chiedo scusa se il mio intervento è stato un po' lungo, ma forse era necessario, com'è necessario proseguire - voglio ribadirlo

anche in percentuale, hanno scelto di accogliere i caduti delle loro Forze armate in forma diversa da quella che noi - con il con il funerale di Stato, con la presenza delle massime autorità e dei Ministri in Parlamento, con la vicinanza vostra e della comunità nazionale, con il minuto di silenzio nei luoghi dove si svolgono attività sportive, con la partecipazione emotiva e sincera di larghissima parte della popolazione civile - abbiamo scelto. Sono orgoglioso di questa mancanza di assuefazione ai lutti: è una specificità italiana, che mi auguro non debba più ripetersi perché mi auguro non ci siano più lutti. Ma quanto avvenuto fino ad oggi ci fa capire come il rapporto tra le forze politiche, le istituzioni, i cittadini e le Forze armate sia un rapporto ormai corretto, di chi comprende che le Forze armate, quei ragazzi e quelle ragazze che sono vere eccellenze dell'Italia, stanno svolgendo il loro compito: sicuramente perché è la loro professione, certamente perché hanno coraggio da vendere e perché sanno di essere preparati per quel compito, ma anche perché sono spinti dalla motivazione più limpida, più vera, più nobile e più alta, quella di servire la nostra Patria in Italia e nei luoghi lontani dai nostri confini. A loro rinnoviamo insieme il nostro grazie e il nostro abbraccio.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innanzitutto desidero associarmi al dolore per i quattro alpini caduti; esprimo le più sincere condoglianze alle famiglie e al 7° Reggimento della Brigata Julia. Desidero anche associarmi alle parole di apprezzamento che lei, signor Ministro, ha voluto esprimere rispetto alla professionalità, alla dedizione e al comportamento delle nostre Forze armate: le condivido. Detto questo, signor Ministro, lei sicuramente ricorderà che i soldati sovietici dell'Armata Rossa, impantanata per dieci anni in Afghanistan, chiamarono i *mujaheddin dushy,* che in russo vuol dire fantasma; già allora avevano capito come, in realtà, si trattasse di una situazione totalmente non convenzionale

chiunque pensi ancora ad una vittoria militare in Afghanistan sia completamente fuori strada; ormai credo di non essere più sola a sostenere questa tesi. Da questo punto di vista, conoscendo un po' la zona, francamente non ricordo né snodi ferroviari, né grandi ponti, né depositi di armi che possano essere fiaccati con bombe, più o meno intelligenti, da 10.000 metri. metri. L'utilità delle bombe, più o meno intelligenti, dunque mi sfugge. Lei ha parlato della protezione dei nostri militari e dei nostri convogli e, giustamente, ha detto che la cosa più importante è l'interrelazione con le popolazioni locali: questa è la nostra «protezione». Rimane il fatto che sembra, non a noi ma in generale, che si faccia e si voglia fare esattamente l'opposto.

Questa non è l'interrelazione con le popolazioni che serve anche per la protezione dei nostri civili. Lasciamo quindi da parte velleità

sostengo da sempre che, non essendoci soluzione militare, l'unica è una soluzione regionale, perché, tra le varie cose, questo Paese è anche circondato da vicini malevoli: un Pakistan che fa il triplo gioco, un Iran che non si capisce bene, eccetera.

Mi auguro che questa sia la soluzione politica verso cui ci si avvii con qualche determinazione

nei confronti dei quattro nostri giovani concittadini: Gianmarco Manca, Marco Pedone, Sebastiano Ville, Francesco Vannozzi, che hanno fatto il loro dovere fino in fondo, fino a rimetterci la vita, a lasciare le loro famiglie nel pianto di un dolore disperato. Loro hanno fatto il loro dovere: ora noi dobbiamo fare il nostro.

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;»

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». I nostri soldati, la nostra bandiera non sono in Afghanistan per fare la guerra, cioè per offendere la libertà di altri popoli o anche solo per risolvere con le armi una controversia internazionale: la Costituzione ce lo vieterebbe e il Presidente della Repubblica, che della Costituzione è rigoroso garante, ce lo impedirebbe. I nostri soldati, la nostra bandiera, sono in Afghanistan per promuovere, se ne saremo capaci, attraverso un misurato e proporzionato uso della forza armata, un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Gli uomini e le donne in divisa che in Afghanistan fanno ogni giorno il loro dovere, rischiando la vita, hanno il diritto di nutrire la certezza di essere lì per questo, per promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, e noi abbiamo il dovere di dimostrare che è così, che loro sono lì per questo e che esiste la ragionevole speranza che questa intenzione possa tradursi in realtà. Altrimenti, dovremmo con onestà riconoscerci tutti nello sfogo del caporal maggiore Luca Cornacchia, il commilitone più fortunato, che è stato solo ferito e al quale mandiamo gli auguri più cordiali per la sua salute. «Mi sono rotto dell'Afghanistan» - ha scritto su Facebook - «non ci capisco niente». Capirci qualcosa è indispensabile per restare lì, sotto il fuoco della guerriglia - lei ha raccontato con particolari, e le siamo grati per questo, di una vera e propria battaglia: non di

non può, non deve significare abbandonare il complesso e faticoso equilibrio di valori e principi ai quali la Costituzione ci richiama; non può significare mollare i freni della ragione e della coscienza, del diritto e della politica e abbattere il senso del limite che impedisce al misurato uso della forza di diventare violenza, quasi non ci fosse tra la pace e la guerra quell'ambigua, difficile e pure preziosa terra di mezzo che è appunto l'uso della forza per promuovere e per conquistare la pace. Negli Stati Uniti, come in Italia, il presidente Obama è fatto oggetto di dure critiche, di attacchi polemici per il suo fermo proposito di muoversi lungo questa terra di mezzo. Lo attaccano i pacifisti, che dicono che è come Bush, lo attaccano i guerrafondai, che lo accusano di essere un soldato riluttante. Noi, signor Presidente, signor Ministro, stiamo con il presidente Obama perché stiamo con la nostra Costituzione, che del resto è anche un po' figlia di quella americana.

vanno guardate dal popolo in un Paese democratico «con guardinga condiscendenza verso un male inevitabile». Sarà per questo che noi italiani, forse noi europei, sentiamo il presidente Obama così vicino, (lei ha detto giustamente e correttamente che c'è stata una svolta nella conduzione della missione in Afghanistan) proprio perché è un soldato riluttante;

mi diceva che avrebbe considerato una sconfitta personale essere costretto a sparare anche un solo colpo. Questo ci rende diversi dagli americani, aggiunse, ma è l'unica strada possibile per conquistare le menti e i cuori degli iracheni. Lei ci ha detto oggi che gli americani sono diventati un po' più italiani da questo punto di vista (forse commenterebbe così il generale della Folgore). Gli americani chiamano il metodo di quel generale della Folgore *soft power*. Obama ha rimesso al centro della strategia politica americana il *soft power*, anche perché il suo predecessore Bush ha involontariamente dimostrato che che l'*hard power*, cioè la potenza dura delle armi, da sola non può tutto e che neanche la superpotenza è onnipotente; anzi l'illusione dell'onnipotenza della superpotenza ci ha consegnato un'America più debole ed un mondo più multipolare, nel quale nessuno, neanche gli Stati Uniti d'America e neanche l'Occidente tutto insieme, può più imporre agli altri la propria volontà. Neppure la lotta al terrorismo di Al Qaeda e al fondamentalismo islamico può essere coronata da successo se non diventa un obiettivo di tutta la comunità internazionale, e del mondo arabo islamico in primo luogo, come fu all'inizio in Afghanistan dopo l'11 settembre e come non è stato invece dopo l'Iraq. Noi vogliamo che l'Italia cammini lungo questa stretta terra di mezzo a fianco dei nostri alleati, del presidente Obama e degli altri europei. La scorsa settimana il ministro della difesa del Governo Zapatero Carme Chacón, in una lunga intervista a «El País», ha affermato che «in Afghanistan il nostro impegno è raggiungere gli obiettivi che l'arrivo di Obama ha permesso di plasmare, in una nuova strategia che la Spagna chiedeva da tempo.

come abbiamo sentito anche dalle sue parole, signor Ministro - un lento e graduale disimpegno che procederà insieme al graduale trasferimento alle Forze armate e alla polizia afgana del controllo del territorio. La Chacón ritiene che entro il 2011 si possano trasferire alle autorità afgane l'aeroporto di Kabul, territori al Nord e al Centro del Paese e - come ci ha riferito anche lei, signor Ministro - una parte significativa della provincia di Herat. Il disimpegno e il trasferimento agli afgani presuppongono il successo di tre azioni parallele: sul piano militare, la difesa e la conquista, non di tutto il territorio afgano (al riguardo poco fa la presidente Bonino ha parole di assoluto buonsenso, perché neanche i sovietici riuscirono a controllare tutto il territorio afgano, con molti più soldati e, peraltro, si calcola che ci vorrebbe almeno mezzo milione di uomini per controllare davvero tutto il territorio afgano, e forse anche in quel caso resterebbero dei dubbi),

Sul piano politico il successo del negoziato con quelli che in modo semplicistico chiamiamo i talebani moderati, che sono in effetti i *pashtun* afgani e pakistani come aveva chiesto l'allora ministro degli esteri britannico David Miliband - con il coinvolgimento delle potenze asiatiche, a cominciare dal Pakistan, ma senza dimenticare l'India, la Russia, la Cina, la Turchia e lo stesso Iran. È una strategia complessa, ma chiara, nella quale l'Italia deve fare la sua parte, non aumentando le bombe, signor Ministro, che rischiano di moltiplicare le vittime civili senza conquistare il controllo del territorio. non a caso Obama ha drasticamente ridotto il ricorso all'arma aerea e ha potenziato le truppe di terra; non a caso l'Amministrazione americana e gli alleati ci chiedono non bombardieri ma istruttori, in particolare dell'Arma dei carabinieri. Noi chiediamo al Governo di muoversi in tale direzione, certi che questa sia la strada giusta, l'unica per la quale abbia un senso ricorrere alla grande professionalità, all'umanità, al coraggio e al senso del dovere di cui i nostri soldati in Afghanistan, come nelle altre missioni all'estero, danno prova ogni giorno.

sono forze irresponsabili che non hanno cura dei nostri soldati e sono degne della massima riprovazione. Noi rivendichiamo, con la massima serietà e determinazione, il sostegno ai soldati impegnati in quel teatro di guerra: è un sostegno convinto, c'è dell'affetto. Lo dico in maniera che potrà sembrare sentimentale: il nostro Gruppo si occupa intensamente della cura e della sopravvivenza dei soldati impegnati in quel teatro di guerra.

il disfattismo richiama antiche memorie: chi non sta in prima fila a difendere la Patria è disfattista e la mette in pericolo.

il ruolo infamante di disfattisti è la stessa che considera 14.000 civili degli sventurati effetti collaterali. Il Ministro rivendica che noi non abbiamo mai causato morti. Ma i nostri soldati, sui nostri mezzi, stanno in un teatro di guerra dove i principali alleati hanno sistematicamente prodotto, con bombardamenti e mitragliamenti dissennati, colpi dall'alto da aerei senza guida, la morte di 14.000 civili. Noi, in quanto alleati, condividiamo - volendo o non volendo - questo segno fortissimo, che impedisce alla radice la costruzione di un clima di confidenza con la popolazione così colpita.

L'intervento in Iraq nasceva da una operazione di falsificazione sistematica che ha avuto origine in Italia sulla famosa questione - che è una "balla" totale - delle armi di distruzione di massa. In Iraq non c'era il terrorismo: il terrorismo in Iraq è arrivato dopo l'intervento; in Afghanistan non c'era il terrorismo, vi è arrivato dopo l'intervento.

dei guerriglieri identificati delle cellule di Al Qaeda, non ci troverete un afgano. Su circa 50.000 guerriglieri censiti dalla CIA, solo 359 sono stranieri e non appartengono alla *jihad*. Quindi, il teorema per cui l'Afghanistan è il nucleo generatore di una offensiva terroristica è completamente falso. Al contrario, la nostra operazione di *peace-keeping (peace-keeping* che viene esercitato con l'arte della guerra, in un teatro di guerra) si sostanza nell'appoggio indiscriminato ad uno dei regimi più corrotti, ad un Governo corrotto, minato da scandali bancari, da innumerevoli conflitti di interesse, da legami tra politica e criminalità

Ricordo di passaggio che il deprecatissimo - giustamente deprecatissimo - Mullah Omar, nel 2000, quando i talebani controllavano il territorio, aveva portato la produzione dell'oppio quasi a zero. Avrà avuto i suoi motivi, ma ciò che va rimarcato è che tutto quello che vediamo oggi come terrorismo è spesso un terrorismo contro un esercito anonimo di robot,

parte. Questa situazione imbarazzante di appoggio ad un regime corrotto e l'impegno in una lotta contro il terrorismo sarebbero giustificati dalla logica che ho sentito più volte ripetere anche in quest'Aula: combattiamo lì per non farli arrivare qui.

Intanto, c'è da provare che potrebbero arrivare qui e c'è da provare il fatto che davvero li combattiamo lì. In realtà lì, nel teatro di guerra afgano, noi stiamo costruendo le condizioni della crescita di un nuovo tipo di terrorismo e di una nuova ondata di terrorismo, sicuramente almeno in quella regione.

alla perfezione da una recentissima intervista del generale Fabio Mini, che non è un pericoloso bolscevico, ma un ex comandante NATO.

quando non ci siamo riusciti negli anni precedenti. Per questo diciamo che bisogna sostenere i nostri soldati riportandoli fuori dal teatro di guerra.

abbiamo perso tragicamente quattro nostri giovani, quattro alpini. Esprimo il cordoglio sentito alle famiglie da parte della Lega Nord, Gruppo che rappresento, e anche i migliori auguri al commilitone ferito. Il cordoglio è anche personale, come bellunese, essendo sindaco di Feltre, luogo dove ha sede il 7° Reggimento Alpini.

Apprezziamo comunque l'impegno del Governo per un programma certo di rientro a partire già dal 2011 concordato con i nostri alleati. Ho chiesto di intervenire, signora Presidente, poiché gli alpini uccisi appartenevano al glorioso battaglione Feltre, che porta il nome della mia città: Battaglione del 7° Reggimento Alpini della Brigata Julia. La città di Feltre ha dato la cittadinanza onoraria agli alpini per i loro meriti, prima di tutto umani, e per il loro amore e protezione della loro terra. Ieri è stato per la città lutto pubblico. Struggenti sono state, durante la solenne messa in Santa Maria degli Angeli, la «Preghiera dell'alpino» ed il canto «Signore delle cime». Ancora più struggenti se riflettiamo sui versi e sull'ambiente descritto e paragoniamo questo al Paese lontano ove sono stati barbaramente uccisi i nostri alpini: deserto, sabbia, terreni aridi a fronte di boschi ed alti prati. Solo le nude rocce in entrambi. La cittadinanza è stata data anche per far sentire a casa loro tutti quei ragazzi, ed ora anche ragazze, che da più parti del Paese arrivano nella nostra montagna. In passato, noi siamo stati terra di elevata emigrazione, per portare sviluppo economico alle zone di origine e di approdo. Vedo similmente questi nostri militari - ma qui parliamo di un bene superiore ed intangibile, la pace e la sicurezza in terre lontane e difficili, ma così anche il mantenimento di pace e sicurezza nel nostro Paese e tra le Nazioni. Sono morti; noi con rispetto diciamo che sono andati avanti per valori ed ideali che troppo spesso passano in secondo piano (e vogliamo onorare le giovani vittime ricordando il motto del 7° Reggimento Alpini**,** *ad excelsa tendo*), che hanno vissuto in modo veramente totale.

pur consapevole dell'impossibilità di attenuare il loro dolore, esprimo innanzitutto ai familiari dei militari caduti un profondo sentimento di cordoglio, e al militare ferito un augurio di pronta guarigione. Come in altre tragiche circostanze, la morte di connazionali in Afghanistan suscita interrogativi sulla presenza dell'Italia in quelle aree di crisi. Da alcune parti si evoca in particolare la necessità di un immediato rientro in Patria dei nostri soldati, perché parteciperebbero ad una missione di guerra e non ad un'operazione di stabilizzazione. Va sottolineato innanzitutto che l'Italia non ha dichiarato guerra ad alcuno, ma è in Afghanistan a seguito di numerose risoluzioni dell'ONU, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Va ricordato, altresì che le operazioni di pace, quelle a cui i nostri soldati partecipano da oltre 30 anni, sempre su mandato dell'ONU, assumono aspetti diversificati, in relazione a comportamenti di chi si oppone a questo processo di stabilizzazione. Sarebbe auspicabile evidentemente uno sviluppo pacifico delle missioni per la pace, ma non sempre è possibile ottenere questo risultato. Quello che deve essere posto a base delle valutazioni in merito alla permanenza o meno, è la sussistenza delle condizioni che hanno indotto l'ONU ad avviare le operazioni. In Afghanistan non credo che possano esserci dubbi al riguardo. C'è ancora una forte opposizione armata al processo di stabilizzazione, la presenza di terroristi nelle zone tribali tra l'Afghanistan, il Pakistan, il Waziristan e nella valle di Swat, rende certo un loro controllo di tutta l'area in caso di disimpegno anzitempo della comunità internazionale. Le forze di sicurezza afgane ancora non sono in grado di garantire autonomamente la sicurezza del territorio. A queste considerazioni c'è da aggiungere il fatto che l'Italia ha assunto impegni precisi nei confronti dell'ONU, della NATO e dell'UE ed è chiamata a rispettare quegli impegni. Un altro interrogativo emerge in queste tragiche circostanze; come si debba fare per garantire la sicurezza dei militari che operano sul territorio. Al riguardo, signor Ministro, ricordo che più di anno fa mi trovai insieme a lei in Afghanistan, subito dopo la morte di un altro soldato italiano. Apprezzai in quella circostanza la decisione che lei prese di non dotare i nostri aerei di bombe ed apprezzai ancora di più le ragioni di tale decisione: le forze italiane non potevano correre il rischio di causare, per errore nell'impiego delle bombe o per imperscrutabile fatalità, sempre possibile, vittime civili; le forze italiane non potevano correre il rischio di dissipare, per errore per imperscrutabile fatalità, il consenso faticosamente acquisito con la loro opera umanitaria. Mi auguro sinceramente che lei voglia confermare quella decisione, anche alla luce delle seguenti considerazioni. Innanzitutto, la paventata ma possibile diminuzione del consenso della popolazione nei confronti dei nostri soldati, in caso di errore o di fatalità, comporterebbe purtroppo un aumento dei rischi di attacco proprio contro quei nostri soldati, a causa della probabile maggiore connivenza che si creerebbe tra l'insorgenza e frange della popolazione delusa. La seconda considerazione si basa su una domanda: ma è opportuno prevedere l'impiego delle bombe sui velivoli nel momento in cui si cerca di applicare la strategia del presidente Obama, contraria ai bombardamenti aerei per evitare i danni collaterali che tante difficoltà hanno creato alla missione e alle Nazioni che sono rimaste coinvolte in quegli eventi?

confermare la decisione già assunta in quella circostanza, garantendo, come ha detto di voler fare, la sicurezza dei nostri uomini attraverso un impiego massiccio - quello sì degli elicotteri, che possono seguire da vicino il movimento dei nostri uomini, attraverso i disturbatori elettronici che possono neutralizzare l'utilizzo delle bombe e infine attraverso l'impiego dei Predator che potranno evidentemente scoprire in anticipo la presenza dell'insorgenza.

e forse non abbiamo la possibilità di avere la dovuta serenità nel giudicare la nostra partecipazione alle suddette missioni, che costituiscono lo strumento vero ed efficace del nostro contributo alla pace. prima di entrare nel merito, desidero anch'io tributare la mia riconoscenza nei confronti dei nostri caduti, non solo dei quattro giovani morti e del soldato ferito, ma anche di tutti i nostri caduti, ed esprimere grande gratitudine nei confronti della lunga linea di centinaia di migliaia di nostri uomini e donne che stanno partecipando a questa operazione che vede l'Italia dignitosamente impegnata nella lotta contro chi vuole sovvertire la pace e lo sviluppo pacifico.

il migliore strumento per attaccare alla radice la minaccia terroristica. auspica un immediato ritorno, a chi critica la nostra presenza, quale sarebbe l'alternativa che propone, perché ancora non l'ho capito. Supponiamo che ci ritiriamo, che le forze alleate si ritirino perché hanno subito tutte quelle perdite: e allora? Ridiamo il Governo ai talebani;

non si risponde alle due risoluzioni delle Nazioni Unite che ordinavano ai talebani di consegnare Bin Laden alla Corte internazionale:

Credo che, se si vuole discutere della nostra presenza, occorra discutere dell'importanza che ha questo strumento di politica estera nelle mani del nostro Governo, del nostro Governo, della presenza corretta e onesta dell'Italia nei confronti delle richieste delle Nazioni Unite, degli impegni della NATO, del desiderio di pace, del desiderio di ristabilire la situazione in Afghanistan, Paese nel quale la soluzione politica alla quale fate riferimento - e non è una novità - era già stata delineata dalle Nazioni Unite. Cari signori,

i santuari pakistani non hanno consentito di eliminare i talebani, perché, se questi fossero stati eliminati e fosse stata chiusa la frontiera del Pakistan, a quest'ora avremmo Karzai, avremmo

come le hanno create in Iraq, dove oggi non c'è più un tiranno e ci si avvia ad avere una soluzione democratica, e come normalmente accade. Per quanto attiene al discorso della guerra, per carità di Dio! La guerra non l'abbiamo dichiarata noi, la guerra ce l'hanno dichiarata gli altri. Vi dimenticate la «guerra ai Crociati», gli atti terroristici? Il terrorismo è un mezzo di guerra, non è un'entità: è un modo e un procedimento. E quelli hanno adottato il procedimento per fare la guerra al mondo occidentale e alla stabilità. Entrando nel merito poi delle due domande che si era posto il Ministro, la prima delle quali è quella relativa agli armamenti, è chiaro che nel momento in cui si è deciso di inviare gli AMX non armati la situazione era diversa. Agli inizi impiegavamo dei mezzi in ogni senso molto più leggeri, perché in realtà la minaccia era inferiore. Nel momento in cui si è affrontato con decisione il problema talebano e si è avuta una forte reazione, nel tempo, come ha ricordato il Ministro, la protezione, gli armamenti, la capacità di fuoco, la capacità di reazione, il controllo del territorio da parte delle nostre truppe sono aumentati. credo non sia nemmeno molto corretto auspicare che noi, per l'impiego a fuoco degli aerei, a chiedere, come già è stato ripetutamente chiesto, il supporto degli americani e degli inglesi: siamo lì, ma non impieghiamo gli aerei e quando servono li facciamo impiegare dagli inglesi, così non corriamo il rischio

in copertura da parte dei servizi segreti è già in atto da anni con la parte buona dei talebani; ma se ad un certo punto non si riesce a far sì che costoro costituiscano una maggioranza nell'ambito del complesso talebano, che si rafforza sempre di più se ha successi, anche quel tentativo fallirà, resterà coperto e non verrà mai alla luce. desidero esprimere ancora la solidarietà ai nostri uomini, non solo ai caduti, ma anche alle migliaia che lì hanno operato. Desidero soprattutto inviare un pensiero di grande stima alle famiglie di questi nostri soldati. Non mi citate quello che scrive su *Facebook*, uno dei tanti. Citatemi tutte le manifestazioni magnifiche che, da quando abbiamo avuto dei caduti, hanno dato le famiglie, le dimostrazioni di orgoglio, la lettura delle lettere che scrivevano questi ragazzi. ragazzi. Debbo dire che questi tristi episodi hanno dato un'idea della sostanza etica e morale del nostro Paese, esemplare in tutto il mondo. Io cerco di ispirarmi a questa dignità e a quest'orgoglio.

ogni volta che si verificano questi tragici eventi siamo costretti a tenere anche la contabilità dei nostri morti in Afghanistan: sono in tutto 33. Signor Ministro, abbiamo apprezzato le sue considerazioni di carattere preliminare sulla natura della nostra missione in Afghanistan, sulla corretta interpretazione del ruolo internazionale del nostro Paese e sulla circostanza che questa, come le altre missioni di pace, siano assolutamente in linea con la la nostra Costituzione e con i principi e le norme che regolano il diritto internazionale. Non è certamente la disputa o la disquisizione in ordine ai termini

il terrorismo internazionale sia un male assoluto, che ha bisogno di forme di contrasto che non sono legate solo alla difesa del nostro territorio in senso stretto.

Non solo dopo questa vicenda, ma per l'evoluzione dei rapporti internazionali e anche della posizione del Governo americano nello scenario di guerra in Afghanistan, oggi si pone il tema di quale debba essere il ruolo dell'Italia, che è stato concepito originariamente, con riferimento a questa missione così come a quella che riguarda l'Iraq, come complementare per la ricostruzione civile

la linea del Governo americano ed anche lo scenario temporale in cui questa missione principale (cioè quella di combattere i talebani) si trova un orizzonte diverso, anche il nostro Paese, che svolge un compito che non è bellico ma di protezione umanitaria, di ricostruzione civile, di assistenza, formazione e costruzione di una parte importante della società civile afgana, si deve interrogare su ciò che deve fare, su come lo deve fare e soprattutto su quale debba essere la linea, non solo di difesa in senso stretto, cioè dell'attività di difesa che noi facciamo in quel territorio, ma la linea di politica estera da seguire. da seguire. Non possiamo certamente esaurire tutto questo in un importantissimo dibattito - e la ringrazio - che si svolge in sede di informativa. Ma è chiaro che vi è la necessità che su questo il Governo con chiarezza formuli una proposta al Parlamento dicendo cosa vuole fare, se vi sono dei cambiamenti anche sotto il profilo delle regole di ingaggio, delle modalità di natura squisitamente militare attraverso cui si esplica la nostra presenza in quel territorio e soprattutto qual è

coinvolti in questa vicenda: dopo l'acquisizione di questi elementi, il Governo potrà formulare una proposta al Parlamento su cui lo stesso sia messo nelle condizioni di poter decidere. Altrimenti animiamo un dibattito che non serve né al Governo, né al Parlamento, né al Paese perché alimenta una confusione che su questi temi non è più possibile. È evidente infatti che, quando un autorevole ex esponente del suo Governo, che oggi è Governatore di una delle Regioni più importanti del nostro Paese, il Veneto, dice che l'Afghanistan è per l'Italia come il Vietnam lo è stato per gli americani si rende conto che tutto questo crea un problema, nel senso che noi vogliamo sapere come e cosa dobbiamo fare lì, per quanto lo dobbiamo fare e in che termini. Lei, molto Lei, molto opportunamente e correttamente, ha detto che le questioni sono due: la prima riguarda la durata della missione, la seconda riguarda la dotazione di mezzi e di risorse e quindi anche le condizioni attraverso cui il nostro contingente opera nella sua missione di pace e ovviamente in condizioni di sicurezza. Quanto alla prima questione è evidente - ripeto

in questa vicenda, cosa si dovrà fare. Ma è altrettanto evidente che a questo vertice, così come alle discussioni di carattere internazionale che nelle prossime settimane e mesi si faranno anche in sede NATO, l'Italia dovrà arrivare preparata e con una propria linea. Noi vorremmo sapere lei lo ha accennato, ma sarebbe opportuno che venisse consacrato in atti ufficiali asseverati dal Parlamento, perché credo che sia anche questa la migliore garanzia per il Governo di avere

meglio di me, avendo noi assunto l'impegno di incrementare il nostro contingente militare a 4.000 unità nelle prossime settimane e poiché tutto questo nasce dalla circostanza di rendere più sicura quindi anche di affrancare il Governo afgano in un momento difficile nella trattativa anche con i talebani, è evidente che in questo periodo l'incremento del nostro contingente

al 2011 della nostra presenza in termini consistenti in quella regione. E poiché comunque questo incremento di contingente determina anche un aumento della nostra attività e della sicurezza del nostro contingente, l'aumento della nostra attività su quel territorio espone obiettivamente a rischi. Lei, con molta franchezza, nella sua introduzione ha detto una cosa ovvia, da alcuni punti di vista, ossia che le condizioni di pericolo nascono dalla situazione che si che si vive ad Herat, che si vive in Afghanistan, e quella è oggettiva; non la possiamo modificare. Possiamo tentare in qualche modo di contenerla e possiamo tentare in qualche modo di tamponarla, ma se noi dicessimo all'opinione pubblica che i nostri militari luoghi a fare una scampagnata credo che non diremmo la verità e faremmo torto anche al dibattito di questa mattina. Allora, è evidente che bisogna anche fare un'operazione verità, che serve a rafforzare il consenso attorno a questa missione, così come vanno rafforzati sempre il consenso e la solidarietà - su questo siamo d'accordo totalmente con lei - del nostro Paese e del Parlamento nei confronti di tutti i militari che sono impegnati in missioni internazionali all'estero. L'altra questione che credo sia estremamente importante è quella della sicurezza. Lei ha avuto modo di chiarire oggi nella sua informativa che non vengono e non saranno cambiate le regole d'ingaggio decise e definite in sede NATO, e quindi noi non cambieremo la modalità attraverso cui svolgiamo la nostra missione in Afghanistan. Credo quindi che a questo punto il tema non sia mettere o non mettere le bombe sugli aerei e consentire agli aerei di bombardare o meno. *(Richiami del

Così com'è avvenuto con i Tornado, non credo che questo sia il tema dirimente, perché se vediamo la stragrande maggioranza degli attentati che sono avvenuti in danno dei nostri militari, sono avvenuti sono avvenuti o con imboscate o con ordigni esplosivi, per cui non penso sia risolutivo ai fini della sicurezza dei nostri militari armare i bombardieri. Ritengo che invece sia opportuno anche su questo immaginare come più complessivamente si garantiscono le condizioni di sicurezza del nostro contingente. Quindi non possiamo, e non potete, neanche alimentare un dibattito surreale su questa vicenda, perché ciò farebbe torto alla serietà della nostra missione; dovreste quindi venire in Parlamento a proporci un percorso, sia sotto il profilo della linea di politica estera che il nostro Governo deve tenere nell'alleanza con gli Stati Uniti, e quindi nel rapporto con il Presidente degli Stati Uniti e con gli altri *partner*, sia con riferimento alle condizioni complessive della presenza dei nostri militari in quel territorio, anche con riguardo alla sicurezza. E va fatto in Parlamento, va fatto qui, con atti concreti, con mozioni, con risoluzioni, su proposte chiare, nette e non propagandistiche del Governo.

«dobbiamo a questi ragazzi infinita riconoscenza per aver sacrificato le loro giovani vite servendo con altruismo e coraggio una causa giusta e facendo onore nel modo più alto al loro e nostro Paese, all'Italia». Sono parole del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, e credo non ci siano parole migliori per esprimere insieme il sentimento di dolore, il sentimento di solidarietà alle famiglie, ma anche il sentimento di fierezza per il comportamento dei nostri soldati, dei nostri caduti: il senso di fierezza per la loro professionalità e per la loro sensibilità. Signor Ministro, le dico subito che abbiamo apprezzato molto l'impostazione che lei ha ritenuto di dare al confronto parlamentare. Riteniamo che questo suo approccio debba essere valorizzato, nel senso che siamo del parere che, in un momento di dolore e di solidarietà,

Riteniamo cioè che ricercare la via della condivisione parlamentare e una comune responsabilità nella fase che si è aperta

quello di rispondere non recuperando un vecchio dibattito che lei - mi permetta, signor

posizionare bene il nostro intervento, la scelta che il nostro Paese ha compiuto, e creare quel clima che consenta di rispondere a questa domanda: quali sono le scelte che bisogna compiere per determinare le migliori condizioni di sicurezza per i nostri soldati?

conseguono e determinano una maggiore sicurezza per i nostri soldati, seppur nella consapevolezza che tutti abbiamo che la risposta, il sì, riguarderebbe solo alcuni casi e solo alcune particolari evenienze, nella consapevolezza che i rischi e anche le vittime sono state causate da condizioni di contesto che non riguardano tanto il tema che lei ha ritenuto di porre in termini tecnici per garantire maggiore sicurezza ai nostri militari. Così come, signor Ministro, sottolineato e ribadito che per quanto ci riguarda la linea non può che essere quella della coerenza con gli impegni sottoscritti in sede NATO, quindi l'esigenza di rapportarsi a decisioni comuni e condivise nel contesto internazionale, io credo che il suo approccio sia responsabile anche rispetto

che forse è inutile indicare date; piuttosto è meglio rafforzare l'idea del processo, del percorso, dell'iniziativa forte, della capacità di armare di più la politica intesa come negoziazione e

con una posizione per quanto ci riguarda probabilmente diversa rispetto all'esito della sua riflessione - che "aggredire" la fonte delle risorse e dei finanziamenti sia una scelta strategica da impostare e rafforzare. anche l'indicazione di processo che lei ha fornito rispetto al ritiro delle truppe ci sembra equilibrata e responsabile e tale da consentire di affrontare correttamente e con responsabilità le questioni che abbiamo di fronte. signor Ministro, il percorso parlamentare che lei ha individuato, sia esso quello del dibattito in Aula o in Commissione, rende questo nostro confronto di oggi una sorta di anteprima rispetto a quel dibattito stesso. Mi auguro, proprio perché sottolineo e ribadisco che condividiamo l'approccio che lei ha ritenuto di utilizzare in questa circostanza così delicata e difficile, che lei stesso contribuisca insieme al Governo, e non solo quindi per la sua responsabilità di Ministro, a sciogliere quei «se» che lei ha posto alla fine del suo intervento.

riguardano la capacità del Governo di dare una risposta rassicurante, tranquillizzante, tale da dimostrare, con profilo strategico, strutturale, continuativo e non episodico, che il Governo accompagna con le risorse e le iniziative necessarie le scelte che intende proporre in sede parlamentare per chiudere la proposta che il Governo ha il dovere di fare per dare conclusione al processo parlamentare che si è aperto con la sua informativa di oggi. Noi rispetto a queste proposte saremo attenti, saremo responsabili, pronti a dare il nostro supporto, a confermare la nostra condivisione, ad esprimere la nostra solidarietà, a determinare cioè tutte quelle condizioni perché davvero si realizzi il suo auspicio che è anche il nostro: far sentire ai militari impegnati la coralità della Patria, la coralità ed il sostegno di tutte le forze politiche e parlamentari.

se si debba parlare (e come e per quando) di ritiro dall'Afghanistan; cosa è più ragionevole immaginare di fare a proposito dei mezzi militari;

rinnovo anche nell'Aula del Senato i sentimenti di gratitudine, di affetto, di vicinanza e soprattutto di grande apprezzamento per quello che i nostri militari hanno fatto e fanno nelle missioni all'estero ed in Afghanistan, con professionalità, con dedizione, con grande capacità operativa e di integrazione con le popolazioni locali, cosa che rende i nostri militari una realtà unica al mondo per affidabilità, qualità del servizio che rendono, serietà. Questo rende più doloroso il sacrificio dei nostri uomini e più grande la nostra responsabilità in questi momenti. riguarda la durata della missione ed il possibile ritiro. Una missione internazionale non può essere né breve, né infinita. Non può essere infinita perché sarebbe una contraddizione insostenibile rispetto alle ragioni stesse della missione, che ben conosciamo. Non può essere breve perché sarebbe incompatibile proprio con la situazione complessa, difficilissima dell'Afghanistan: un territorio dove nei secoli chi, venendo da fuori rispetto alla complessa struttura tribale e all'articolazione dei poteri e agli interessi spesso non trasparenti in campo, campo, vi si è misurato ha pagato prezzi altissimi. Ecco perché la condizione nella quale ci troviamo oggi, che è quella di una presenza massima nella storia delle missioni internazionali in Afghanistan, ha un senso, una ragione. Mai tante truppe (circa 150.000 uomini) sono state presenti in Afghanistan: 30.000 uomini in più di quelli che l'Unione Sovietica aveva schierato al culmine delle sue operazioni militari negli anni Ottanta. Il *timing* per un possibile rientro delle nostre truppe, signor Ministro, non può che essere ovviamente collegato alle decisioni della comunità internazionale e non può che essere coerente con una strategia di lungo termine.

non assistito da deliberazioni delle Nazioni Unite che aveva diviso la comunità internazionale e l'Unione europea, mentre oggi siamo in Afghanistan - chiunque può dissentire, naturalmente - sulla base di un mandato molto largo e di una partecipazione, che origina ovviamente dalla tragedia dell'11 settembre, molto significativa. Colleghi, penso che sarebbe un guaio se un giorno noi dovessimo pentirci di un abbandono prematuro dell'Afghanistan, e i primi a chiederne conto sarebbero i familiari delle vittime e tutta l'opinione pubblica dopo almeno un decennio di impegno e di spese. Ci terrei che il Ministro ascoltasse. Non so se il senatore Gramazio deve parlare delle ASL della Regione Lazio (che fa anche rima), ma forse sì. Vista l'intensità della conversazione, immagino che stiano parlando delle ASL della Regione Lazio.

la politica incoerente che va sotto il nome di «mordi e fuggi» non ha dato buoni risultati. Ed era assolutamente inadeguata l'integrazione delle iniziative per la sicurezza con quelle per la stabilizzazione civile e istituzionale. signora Presidente, un fatto positivo anche nella collaborazione tra le opposizioni e i Governi. Era la posizione del Governo precedente quella di una maggiore integrazione tra attività militari e civili, ed è positivo che l'attuale Governo l'abbia assunta e fatta propria, certamente anche alla luce delle aspettative poste dalla nuova amministrazione americana, che ha "liberato" le energie impegnate in Iraq per concentrarsi sulla crisi afgana. Soprattutto, ha allargato l'orizzonte strategico con riferimento alla regione, al Pakistan, e ad una visione maggiormente integrata. Adesso siamo alla vigilia di tre passaggi: riunione a Roma con Petraeus, Vertice della NATO a novembre, *review* dell'amministrazione americana a dicembre; però è anche vero che dobbiamo prendere alcune decisioni che derivano dal derivano dal fatto che le operazioni in corso accrescono i pericoli per i nostri soldati, non li riducono. La situazione attuale, con i combattimenti a Kandahar, Marjah e nell'Helmand, condotti da truppe americane e britanniche spostano l'area di azione dei talebani verso nord-ovest, lì dove sono i nostri soldati. Il processo di riconciliazione con una parte dei talebani avviato da Karzai fa sì che chi per il momento è fuori dalla trattativa «spari tutte le cartucce»

l'equivoco su una *exit strategy* non ci deve fare dimenticare che oggi siamo in Bosnia e in Kosovo 15 anni dopo l'intervento: non è pensabile che si rimanga in Afghanistan come se quella complessa situazione sia risolvibile in poco tempo.

di tipo aereo anche con gli elicotteri o l'utilizzo dei droni Predator, che hanno una capacità di precisione teleguidata sicuramente significativa. Sono argomenti tecnici sui quali oggi non si pronuncia il Parlamento: lo farà al momento giusto. Io osservo però che dobbiamo mettere in campo tutti i mezzi che tutelino la sicurezza e l'operatività dei nostri soldati. ho apprezzato che il ministro La Russa si ponga, nel contesto di queste decisioni, l'obiettivo di non dividere il Parlamento. È evidente, infatti, che dobbiamo mantenere attorno a questa missione il massimo di unità nel nostro Paese; sarebbe impensabile che si creasse una spaccatura. Signora Presidente, in un Paese serio sulla politica estera si formano le maggioranze,

Un anno fa il generale McChrystal, prima del suo ritiro, ha sostanzialmente affermato che la strategia adottata non permette di vincere.

e ai suoi santuari e si sta contrastando la prospettiva che l'Afghanistan torni ad essere piattaforma logistica per il terrorismo internazionale e le sue reti. Si può affermare che i talebani stanno vincendo in Afghanistan

parola guerra su argomenti come la mafia, la camorra e la droga, noi dell'Italia dei Valori la sottoscriviamo anche oggi stesso, davanti a tutti.

Signor Ministro, faccia le sue considerazioni, ma rifletta sui militari che dicono esattamente l'opposto di quanto ha comunicato lei pochi minuti fa. Lei dice che Herat è stata ormai consegnata e si sono impiegati

Un solo Paese ha avuto la coerenza di capire l'errore, l'Olanda, ma lei non ne ha parlato. Ha parlato solo dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Caro Ministro, non esistono bombe di pace o bombe di guerra. Non esistono morti di pace o morti di guerra. Esistono invece le responsabilità politiche e morali di chi queste bombe e queste morti usa e ha usato. Ministro La Russa, lei ha questa responsabilità, e con lei il Governo Berlusconi. Lei ha questa responsabilità quando propone di dotare di armi micidiali i nostri aerei, imponendo al conflitto afgano l'ultima *escalation* che mancava. Lei ha questa responsabilità quando i nostri ragazzi rientrano in Italia, come ieri, da vittime di una guerra con le armi che non vogliono e che non volevano. Lo hanno scritto più volte - come ha ricordato anche un collega

Lei ha questa responsabilità quando non riconosce che in Afghanistan la guerra si combatte e con inaccettabile irresponsabilità propone di dotarsi di bombe. Forse è con queste che intende costruire gli asili per i bambini afgani o addestrare la polizia di Karzai? Nel nostro Esercito ci sono ragazzi che non trovano più impiego. Sono giovani che devono scegliersi il proprio futuro, tra una mafia mai combattuta da un Governo con alcune persone che lo rappresentano e la povertà. Per sfuggire all'una e all'altra scelgono l'Esercito, sperando forse di imparare nelle missioni all'estero all'estero come si fa la cooperazione allo sviluppo, il sostegno alle popolazioni martoriate dai conflitti, la ricostruzione di logistiche e infrastrutture nei Paesi dilaniati. Al per la sua responsabilità, si trovano senza regole di ingaggio adeguate a cercare di rimanere in piedi sotto il fuoco nemico. Non le elenco i dati perché lo ha già fatto ieri il presidente Di Pietro.

dividerle e a vestirle a lutto, come invece purtroppo è successo. Da quanto tempo l'Italia dei Valori chiede il ritiro del contingente dall'Afghanistan, Ministro? Abbiamo iniziato dal 2009, in una Commissione esteri sorda, quando un Parlamento meno distratto e un Governo meno occupato a farsi gli affari suoi potevano già comprendere che la frase «siamo in guerra» era diventata ormai retorica. Noi siamo la parte che rappresenta l'Italia che non vuole stare in Afghanistan in questo modo. Abbiamo votato contro il rifinanziamento di questa missione, che nel tempo ha cambiato natura, connotati e scopi. Abbiamo votato contro, perché ormai è chiaro che combattere in una guerra tra fazioni non porta risultati, in termini né militari né civili. Abbiamo votato contro perché non si combattono i presunti terroristi in guerra straniera per non farli venire nel nostro Paese in questo modo. Anzi, la storia, purtroppo, ci ha insegnato che i terroristi compiono atti violenti proprio contro quei Paesi che sono in prima fila con le armi e con le bombe. Abbiamo votato contro perché non abbiamo ancora capito quali sono gli interessi celati che ci tengono lì. Signor Ministro, legga quanto ha detto Cecilia Strada, che ci sta tutti i giorni in quei territori, per fare capire a lei che sta in Italia come si vive in quel Paese. E abbiamo votato contro perché non vogliamo leggere l'articolo 11 della Costituzione come lo legge lei, come lo interpreta lei e come lo utilizza lei, come ha utilizzato le parole che il Capo dello Stato non voleva dire in tali termini, e lei le ha utilizzate in un modo che ministro La Russa, quando è venuto in Senato per piangere altri ragazzi morti ammazzati, senza poi riuscire ad impedire che altri se ne dovessero piangere, mi ha detto in modo provocatorio di continuare la lettura dell'articolo 11 della nostra Carta costituzionale dato che le avevo citato solo le prime parole. Ebbene, l'accontento: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». parole, signora Presidente. Vuole forse dirmi, signor Ministro, che tra noi e gli Stati Uniti c'è una condizione di parità? Vuole forse dirmi che limitiamo il nostro potere... Il Senato sta perseguendo quello scopo a Kabul? Signor Ministro, basta con le ipocrisie. Ammettete di aver fatto un grande errore. L'Italia dei Valori non accetta e non accetterà mai il suo modo di intendere la pace. Andiamo via dall'Afghanistan adesso e non a parole. Andiamo via perché già troppo tardi.

e del Gruppo che rappresento alle famiglie dei militari caduti in Afghanistan lo scorso sabato 9 ottobre. È un cordoglio che desidero unire ad un sincero ringraziamento ai nostri ragazzi per tutto quello che hanno fatto in quelle e in altre terre difficili, per decisione del Parlamento. Il grave incidente che ha provocato la perdita dei quattro alpini non rappresenta, purtroppo, un fatto eccezionale nell'attuale contesto afgano. Occorre ricordare, infatti, come in oltre il 60 per cento dei casi i militari siano stati uccisi da ordigni esplosivi artigianali e che rispetto a tale tipo di minaccia esistono pochissime difese. Vorrei altresì manifestare tutto il mio apprezzamento per la tempestività dimostrata dal Ministro della difesa ad accogliere l'invito del Senato a ricostruire l'accaduto perché ha pubblicamente dichiarato di voler ascoltare e recepire il parere delle Commissioni difesa del Senato e della Camera (anche se non è vincolante) per decidere sull'eventualità di equipaggiare in maniera offensiva i nostri aerei di stanza in Afghanistan,

Si è molto parlato nei giorni scorsi, soprattutto a caldo, di come ridurre i rischi che gravano sui soldati italiani e della strategia che sono stati chiamati a realizzare. Ora, però, è il tempo dei ragionamenti ponderati, lucidi e freddi, per stabilire cosa fare nell'immediato futuro. La Lega Nord ha sostenuto e sosterrà lealmente il Governo nelle sue scelte relative alle missioni internazionali di pace: un Governo, che ha onorato sempre, con grande senso di responsabilità e lealtà, i suoi militari, uomini e donne, sparsi nel mondo, impegnati nelle missioni e ha onorato altresì le tre più grandi organizzazioni mondiali - l'ONU, la NATO e l'Unione europea - di cui il nostro Paese fa parte. Chi si aspetta dalla Lega uno strappo o un gesto di rottura su questo delicato aspetto della politica del nostro Paese rimarrà deluso: ci teniamo a sottolinearlo. Questo non vuole dire però che si debba rinunciare a pensare di riportare a casa i nostri uomini, soprattutto di fronte alle difficoltà che si stanno palesando.

come al solito, per distinguersi, mostrano tutta la loro ipocrisia politica. Si tratta di ragionare sulle prospettive delle operazioni e sullo scenario di un impegno graduale, tenendo presente quanto stanno facendo i nostri alleati.

Tutti vorremmo vedere in tempi brevi un Afghanistan stabilizzato, lontano dagli eccessi del fondamentalismo islamico; tutti vogliamo al più presto riportare i nostri militari a casa, invece di guardarli dagli schermi dei nostri televisori a tempo indeterminato, e purtroppo quando tornano in veste di caduti. Tutti saremmo felici di rimpatriare i militari a rischio *combat* nel nostro contingente entro il 2011. Apprezziamo quanto detto da lei, signor Ministro, sull'impegno di far rispettare determinate date, ma siamo anche chiamati ad onorare una responsabilità, e rientra nel concetto di responsabilità rispettare l'impegno che ci siamo assunti quando, nel dicembre 2001, in occasione della Conferenza internazionale di Bonn, gli afgani ci chiesero di aiutarli a ricostruire il loro Paese. Decidemmo di accettare, anche per allontanare la prospettiva del terrorismo dalle nostre terre, ben sapendo che in Afghanistan si trova il vertice di Al Qaeda. Onorare gli impegni assunti con il Governo di Kabul non significa però che ora dal presidente Karzai non si possa chiedere e pretendere qualcosa in cambio. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi la sua amministrazione faccia finalmente quello che è necessario, operando per rendere più efficiente il suo Stato, che latita persino nelle forniture dei servizi più elementari, combattendo la corruzione, nominando funzionari sul territorio, senza per questo ricorrere alle logiche di affiliazione, in modo tale da tagliare finalmente l'erba sotto i piedi ai talebani e a chi li fiancheggia.

questo un valore assoluto e noi riteniamo che in una democrazia non si possa prescindere dal valore assoluto della componente femminile; senza questi passaggi essenziali, infatti, si fallisce, e non c'è prospettiva basata sulla restituzione agli afgani della competenza sulla propria sicurezza nazionale. Ciò che chiediamo a Karzai è di contribuire con coraggio politico al nostro impegno militare; senza questo fattore essenziale, il nostro intervento, occidentale ed italiano, è destinato a rivelarsi inutile e infruttuoso. È bene sottolineare come un ritiro graduale delle forze occidentali in Afghanistan a seguito di un eventuale accordo raggiunto con i talebani storici porrebbe un problema politico sulla gestione della transizione; un eventuale ritorno del mullah Omar a Kabul, anche nel contesto di un governo di coalizione, susciterebbe verosimilmente reazioni molto ostili. Non è quello che ci auguriamo, soprattutto oggi che piangiamo e commemoriamo i nostri caduti. Auspichiamo invece il nostro successo, anche perché da quello dipende la stessa sicurezza delle nostra città: città che siamo riusciti - e non dimentichiamocelo - a proteggere finora più efficacemente dei nostri alleati inglesi e spagnoli. Oggi, come nei trascorsi nove anni, la posizione della Lega Nord non cambia; vogliamo che i nostri soldati possano difendersi al meglio ed avere tutto ciò che è giudicato necessario a questo fine; ad altri, più esperti di noi, rimettiamo il compito di determinare cosa davvero occorre per raggiungere tale obiettivo. In conclusione, signora Presidente, signor Ministro e colleghi, vorrei ribadire che noi siamo e saremo sempre a fianco dei nostri militari, che desideriamo ringraziare ed onorare una volta di più per quanto fanno.

Per quanto riguarda il merito della nostra discussione, devo dire che non convince l'intervento effettuato in quest'Aula questa mattina dal ministro La Russa, che parla di diritto, di dotazioni di armi, lasciando però insoluti i dubbi di partenza di questa vicenda.

soprattutto quando abbiamo assistito in questa legislatura da parte del Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri a una mortificazione ripetuta e continua delle funzioni e del ruolo del Parlamento. Ritengo che due siano gli aspetti fondamentali che invece vanno ribaditi e chiariti. Innanzitutto va chiarita per bene e fino in fondo quale sia la natura della missione,

Il secondo aspetto fondamentale è che noi siamo assolutamente a favore della sicurezza dei soldati, che va garantita in ogni modo. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, mi limito a dire che la proposta delle bombe sugli aerei italiani è assolutamente fuorviante e pericolosa. Già stamattina in quest'Aula il senatore generale Del Vecchio, ma anche altri tecnici tecnici e militari come il generale Tricarico ci hanno ricordato che assolutamente le bombe sugli aerei non servono per la sicurezza dei soldati. Noi abbiamo già elicotteri dotati di mitragliatrici che possono entrare in gioco quando c'è bisogno di sorvoli sulle colonne di blindati ed intervenire secondo le regole d'ingaggio esistenti per rispondere ad eventuali attacchi, oltre che con effetto deterrente. Ricordo inoltre il cambio (non recentissimo, ma comunque recente) della strategia e della politica del Pentagono. La nuova strategia, prima del generale McChrystal e poi di Petraeus, è stata quella di mettere più uomini sul territorio proprio per avere una minore ostilità da parte della popolazione civile

perché bisogna passare dall'impegno militare a un sempre maggiore e possibilmente esclusivo impegno politico e sociale a favore delle popolazioni civili.

Signora Presidente, onorevole Ministro, non tanto tempo fa - è trascorso solo qualche decennio - una parte del mondo si domandò se fosse possibile morire per Danzica. Solo dopo si chiarì quanta incomprensione si condensava in quell'interrogativo. Non ripetiamo lo stesso errore oggi. L'Afghanistan ha rappresentato uno degli snodi più sensibili del passaggio dalla guerra fredda al nuovo Lì, al tempo dell'invasione dell'Unione Sovietica - lo ha ricordato lei, signora Presidente - si ruppe il fronte islamico, con la parte fondamentalista che divenne protagonista della guerriglia antisovietica e gli Stati più secolari che confermarono, invece, un'alleanza storica sorta nel secondo dopoguerra, quando il baathismo passò senza soluzione di continuità dal filohitlerismo al filosovietismo. Implosa l'Unione Sovietica, è venuto meno l'elemento che aveva determinato quella divisione e si è creata un'alleanza dal fortissimo significato antioccidentale. Tanto più forte quanto ci si è sentiti protagonisti dell'abbattimento di uno dei due giganti. Le forze, insomma, si coalizzarono contro l'altro. Non si comprende l'11 settembre, non si comprende la guerra asimmetrica, non si comprende la portata del terrorismo internazionale se non si capisce questa dinamica. E l'Afghanistan - la guerra in Afghanistan - rappresenta l'epicentro di questa trasformazione geopolitica. Certo, nessuno vorrebbe dover morire per l'Afghanistan. Soprattutto non lo vorrebbero i cittadini afgani non coinvolti nella guerriglia, i legittimi cittadini di quello sventurato Paese, che da decadi ormai innumerevoli muoiono a migliaia per il diritto di vivere in pace. Neppure noi italiani, noi europei, noi occidentali vorremmo dover morire per l'Afghanistan. Ma neppure vorremmo dover morire al *World Trade Center* di New York, alla stazione Atocha di Madrid, nella metropolitana di Londra o all'hotel Oberoi di Bombay, o per le strade di Tel Aviv o di Gerusalemme. Eppure questo tragicamente accade, da decenni. Neppure i nostri soldati vorrebbero morire per l'Afghanistan e in Afghanistan, eppure anche questo tragicamente accade, e spesso accade anche avendo avendo perso di vista l'evidenza che ci ha condotto su quelle montagne, tra quei valichi, in quei deserti. La lunga durata della guerra ha reso opachi i suoi scopi e più dolorose le sue perdite. È proprio per questo che l'ultima cosa da fare in queste occasioni è accrescere l'opacità, aumentare la confusione, diffondere l'incertezza. Mentre la miglior cosa da fare è andare alle radici della nostra presenza in quel Paese, ritrovarne le ragioni e guardarle con occhi attenti, e se possibile, asciutti. Siamo tutti stufi dell'Afghanistan, come ha detto in uno sfogo più che comprensibile - lo ha ricordato il senatore Tonini - Luca Cornacchia, il militare ferito nello scontro a fuoco di sabato mattina. Il fatto con cui misurarci però è che l'Afghanistan non è stufo di noi: ha bisogno della nostra presenza per non ricadere in un inferno se possibile ancora peggiore di quello in cui l'ultimo regime talebano lo ha costretto per anni. E noi stessi abbiamo bisogno di quella presenza militare proprio per spostare lì la frontiera più avanzata dello scontro con il terrorismo internazionale e allontanarlo dalla Torre Eiffel, dal Colosseo, dalle nostre case, strade e piazze. E per altri versi il problema è che i talebani, i jihadisti più agguerriti, non sono stufi di noi. Non si accontenterebbero di vederci abbandonare l'Afghanistan umiliati e sconfitti: vogliono la nostra sottomissione, la nostra resa senza condizioni, le nostre bandiere ammainate e le loro a svettare sull'Occidente o su quel che ne rimarrebbe. Una democrazia fa fatica a sopportare perdite per una guerra lontana e difficile. I nostri nemici contano su questo, è il cuore della loro strategia offensiva. Non ci possono battere sul campo, ma ci possono sconfiggere nell'animo, possono renderci stufi, divisi, confusi, irresoluti. Noi qui oggi abbiamo il dovere di resistere, di reggere la sfida, esattamente come fanno i nostri soldati sotto il fuoco dei kalashnikov, in marcia verso gli obiettivi più insidiosi. A loro prima di tutto dobbiamo la nostra unità e la nostra determinazione. Mentre loro sono lì, noi non abbiamo il diritto di essere stufi. Possiamo, anzi dobbiamo, esaminare con freddezza le condizioni oggettive dello scontro in atto. Giudicare se le nostre forze sono adeguate, se le condizioni di sicurezza sono assicurate sono assicurate fino al limite del possibile, se le nostre regole d'ingaggio sono aggiornate, se il Pakistan sia o no un interlocutore leale, se le relazioni con gli alleati siano fluide e persino possiamo immaginare le tappe di una possibile *exit strategy*, concordata e condivisa. Il Ministro ci ha chiesto un aiuto, in Commissione da noi non verrà meno questo aiuto. Non c'è eresia in tutto questo. Solo mi insospettisce e un po' mi amareggia che questi temi, pure cruciali, ci troviamo sempre e solo ad affrontarli sull'onda dei lutti e delle polemiche. Improvvisamente diventiamo tutti esperti di tecniche militari, di contro-insorgenza, di sistemi d'arma, di bombe e di missili, come se la guerra in Afghanistan fosse un dato intermittente, che si accende e si spegne solo rispetto alla nostra sensibilità o, peggio, alla nostra inclinazione politica. Nessuno ha risposte precise sul futuro della missione NATO in Afghanistan. Lo stesso Obama, che ho tante volte sentito richiamare in quest'Aula, e i vertici del Pentagono forniscono risposte diverse, hanno punti di vista discordanti, spesso sembrano impantanati nelle dispute. Anche la NATO va avanti per tentativi, per ipotesi, per approssimazioni. Lo dico perché ad un certo punto è sembrato che il Governo italiano fosse privo di lucidità e di strategia.

I nostri vertici militari sul campo si sono guadagnati la migliore reputazione e sono considerati un modello di comportamento, di dedizione e di impegno. Siamo oggi nelle condizioni di aver diritto di parola sulla scena internazionale, di proporre le nostre idee e le nostre soluzioni, sapendo che verrebbero prese sul serio. Ma proprio per questo non troveremo risposte adeguate alle necessità del conflitto se andiamo a cercarle nel risentimento, nello scontro o nella strumentalizzazione. Il Governo, la maggioranza, l'intero Parlamento hanno il diritto di riflettere su un impegno così gravido di costi e di dolori. Ma hanno il dovere di non lasciarsi sopraffare dalla facile retorica del «torniamo a casa», perché altrimenti, alla lunga, a forza di retrocedere, potrebbe non esserci più una casa dove tornare.

per quale motivo l'UEFA non abbia avuto il coraggio di sospendere la partita e la decisione sia dovuta toccare al povero arbitro, che fa parte di una categoria spesso maltrattata, ma che in questa occasione ha avuto il coraggio di fare quello che altri non hanno fatto. fatto. Ci sono aspetti che restano oscuri e sui quali è necessario avere un chiarimento. Chiedo quindi, anche a nome dei colleghi, se il Governo può venire in Aula a riferire sui fatti di ieri sera, che ritengo estremamente gravi.

Ribadisco ancora una volta che inerisce ad un contenzioso tra la Cofiloc spa, un'azienda della Provincia di Treviso, e l'Agenzia delle entrate di Treviso.

Mi sembra assurdo che soltanto un'Agenzia delle entrate, specificatamente quella di Treviso dove abito, applichi un principio assolutamente difforme da quanto previsto dalla normativa generale,

voglio ricordare che mentre i mercati continuano a ballare, il renminbi tiene col fiato sospeso il mondo per la sua mancata rivalutazione (per non dire poi che in Cina ci sono anche problemi di diritti umani), noi da oltre 100 giorni siamo senza il Presidente della CONSOB, la Commissione nazionale per le società e la borsa. Ed è un fatto molto, molto grave, tenendo conto che proprio ieri il presidente dell'ABI e del Monte dei Paschi di Siena Mussari ha affermato che la non regolazione dei mercati produce dei danni. Quindi, chi dovrebbe regolare il mercato è anche una CONSOB efficiente. Su 5 commissari ce ne sono 3: uno si è dimesso per andare, com'è noto, a garantire gli interessi di Caltagirone all'interno del consiglio di amministrazione dell'ACEA. dell'ACEA. Ancora una volta chiedo che si venga a riferire su questi litigi che non fanno nominare il consiglio di amministrazione della CONSOB. il presidente Mussari ha detto che i banchieri che sbagliano vanno in galera. Voglio anche richiamare l'attenzione sul fatto che torna la speculazione. Lo ha detto anche il ministro dell'economia Tremonti questo fine settimana in occasione di un vertice internazionale. La speculazione è anche data del ritorno dei *junk bond*: le obbligazioni spazzatura

Bisogna nominare il Presidente della CONSOB. La CONSOB deve essere messa in grado, anche per riparare ai gravissimi errori del passato, di operare nella pienezza dei suoi poteri, anche perché questo signor presidente vicario viene dalle banche, e certamente non può tutelare i diritti dei risparmiatori e del mercato. Quindi - la ringrazio ancora una volta, signora Presidente

per la quale è stata già avanzata dalla Presidenza una richiesta di risposta in tempi brevi, che ancora sto aspettando. Ho avuto dal ministro Vito segnali che la richiesta del Presidente è arrivata, ma la risposta non giunge. Sono costretta anch'io, alla fine di ogni seduta, a ripetere questa prece, perché quella gente ha bisogno che il Governo mantenga gli impegni presi. finestra"). La Presidenza farà tutti gli accertamenti del caso, ma è indubbio che il problema si pone in termini di strumenti di